Vi prego di votare perché sto per dichiarare chiusa la votazione.

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

Credo stia sfuggendo a questa Assemblea un fatto molto importante, l'estensione di questo scudo fiscale alle società estere controllate e partecipate comporta una vera e propria amnistia per una serie di reati. Chiunque abbia seguito negli ultimi tempi le cronache giudiziarie

come la frode fiscale o il falso in bilancio con una maggioranza semplice attraverso una legge ordinaria, quando la Costituzione prevede che per qualsiasi forma di amnistia

Se pensiamo che effettivamente si possano attuare a cuor leggero queste amnistie vuol dire che legittimiamo in Italia la frode fiscale e il falso in bilancio, con una legge ordinaria. Ma questa è solo una delle questioni che riguardano questo articolo. Un'altra questione molto importante è quella relativa al riciclaggio.

in questo modo si favorisce chiaramente il riciclaggio. Mi chiedo allora: vi siete posti il problema di favorire il riciclaggio e la criminalità organizzata? Vi siete posti il problema che in questo momento, visto che è stato dato parere favorevole dalla relatrice e dal Governo, state concedendo un'amnistia per reati gravissimi?

come il mondo, perché furono inventati da Sindona e poi sono andati via via evolvendosi: e si potrebbero fare esempi infiniti su questo modo di accumulare capitali all'estero e di fare falso in bilancio in Italia attraverso società collegate

È ora che ci guardiamo in faccia tranquillamente e ci chiediamo: vogliamo che il nostro continui ad essere un Paese ad enorme evasione fiscale?

e per dare un aiuto alle famiglie in difficoltà e a coloro che adesso soffrono enormemente per la riduzione delle ore di lavoro e per la riduzione dell'occupazione.

con queste norme favorite il riciclaggio del denaro. Non lo dite più, per favore! Non vi vantate di essere quelli che fanno una lotta seria alla criminalità organizzata; non vi vantate di fare la lotta all'evasione fiscale, e non date cifre che non esistono da nessuna parte.

Se volete farlo fate pure, accomodatevi, ma non avrete mai il consenso di questo Partito Democratico! Signor Presidente, non voglio fare polemica, ma mi permetto di sottolineare un aspetto che riguarda il metodo. Stiamo esaminando un decreto‑legge che ha lo scopo mirato di correggerne uno precedente. Peraltro,

che credo sia inopportuna sotto il profilo del metodo, a prescindere dal merito della questione. Infatti, l'idea di un decreto correttivo - che riguardava, ad esempio, le parti relative alla giurisdizione della Corte dei conti, alla società Stretto di Messina, ai Commissari di Governo e ad alcune altre questioni relative al Ministero dell'ambiente - era ampiamente condivisa e quindi avrebbe garantito

oggettivamente e soggettivamente la portata di tale disposizione. Oggettivamente perché, come è stato ricordato, avete introdotto la non punibilità di una serie di reati societari, a cominciare dal falso in bilancio

di contrasto al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata, e quindi a quella criminalità che si occupa ed esercita le proprie attività prevalentemente attraverso la criminalità finanziaria.

nel dibattito che, anche in Senato, abbiamo fatto sull'uso e l'abuso della decretazione d'urgenza. Va considerato che in ogni decreto-legge, indipendentemente dall'omogeneità della materia trattata, avete inserito in sede di conversione tutta una serie di norme che hanno fatto insorgere il Capo dello Stato (ciò è accaduto anche con riguardo alla vicenda del pacchetto sicurezza) che ha voluto sottolineare la necessità di non esagerare nel percorso di formazione delle leggi e, quindi, di garantire al Parlamento la possibilità di esaminare con chiarezza e in approfondita le disposizioni che si devono approvare. Tutto ciò con l'emendamento 1.3500 è saltato. Infatti, in un decreto correttivo di un precedente decreto, che già era una forzatura sul piano istituzionale, avete inserito, in sede di conversione, una norma che ha di fatto stravolto la disciplina sullo scudo fiscale,

con queste furbizie in forza delle quali il Governo non sa nulla e sono alcuni colleghi della maggioranza che in sede di conversione del decreto presentano gli emendamenti. A queste considerazioni aggiungo che tutta la normativa

è una dichiarazione di voto per consegnare agli atti la portata di questo ennesimo regalo che fate agli evasori: il terzo riciclaggio di Stato varato ancora una volta dal ministro dell'economia Tremonti, che prometteva sempre che sarebbe stato l'ultimo. questo scudo esclude l'obbligo di segnalazione ai fini dell'antiriciclaggio in capo agli intermediari finanziari, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, che evidentemente spaventa molti possibili fruitori dello scudo e che minacciava di ridurre il gettito. L'esclusione ad ogni effetto della punibilità riguarda fattispecie come: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, occultamento o distruzione di documento; falsità materiale commessa dal privato; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; falsità in registri e notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso; soppressione; distruzione e occultamento di atti veri; falsità in documenti informatici e copie autentiche in luogo di originali mancanti; false comunicazioni sociali; false comunicazioni in danno della società, dei soci e dei creditori; falso in prospetto. Non si capisce, cioè, cosa resta dopo questo scudo.

con questo scudo, per incassare forse 5 miliardi su 100 lo Stato è disposto a regalarne 10 a pochissime banche. In Inghilterra - l'ho ricordato anche ieri - evasori e riciclatori su 100 sterline ne devono spendere 51. Rivolgo un ulteriore invito a riflettere, però sappiamo che è difficile far ragionare questo Governo e questa maggioranza sull'etica della responsabilità e sulla legalità. Presidente, non se ne dispiaccia la mia Capogruppo, ma contrariamente alle indicazioni non parteciperò al voto sull'emendamento 1.3500/1. Voglio ricordare ai colleghi che qualche anno fa un avvocato di nome Giorgio Ambrosoli, a Milano, scoprì che una cosiddetta banca d'affari, guidata da un personaggio che si chiamava Michele Sindona,

L'ha già detto il senatore D'Ambrosio. In quest'Aula abbiamo varato molti provvedimenti e alcuni esponenti della maggioranza si sono anche piccati di fare con le norme e con il loro voto una dura battaglia contro la criminalità. Siamo d'accordo; siamo stati concordi su questo, ma adesso devono spiegare a quest'Aula penso che tutti dobbiamo stare molto attenti - e al Paese l'attacco in atto ad un punto fondamentale: stiamo favorendo il riciclaggio. Sappiamo che la criminalità non si contrasta soltanto con il carcere duro o con qualche altra norma; bisogna attaccare al cuore, e il cuore sono le attività economiche illecite. Se su questo c'è omertà, c'è grande responsabilità di questa Aula e delle forze politiche di fronte alla Nazione.

in quanto la Commissione giustizia non l'ha mai vagliato. È stato presentato in Aula operando un intervento pesante su una complessità di reati che vengono amnistiati ed indultati: infatti, mentre il provvedimento precedente stabiliva che questi elementi non possono essere valutati autonomamente, ma si può arrivare alla punibilità attraverso altri accertamenti, con il presente

e i poteri che deve avere la Commissione giustizia in materie così delicate.

sarebbe sufficiente non argomentare dicendo solo che questo emendamento presentato così provvidenzialmente dal senatore Fleres è una vergogna ed uno scandalo! So anche che le ragioni giuridiche e politiche - laddove la politica normalmente nelle democrazie avanzate viene innervata dai princìpi che riguardano da una parte la legalità e dall'altra parte, come ricordava il senatore D'Ambrosio, l'etica pubblica le argomentazioni che svolgerò non troveranno un grande ascolto da parte dei colleghi della maggioranza, i quali non hanno esitato, per mano del senatore Fleres, a rompere una delicata intesa istituzionale, un delicato equilibrio che, sia pure per vie molto perigliose, come ci ricordava il presidente D'Alia, era arrivato alla confezione di un decreto-legge correttivo di un decreto-legge approvato con un voto di fiducia, che a sua volta correggeva un testo precedente. Però, alcune considerazioni vanno comunque fatte, se non altro perché mentre qui, con l'insofferenza che è tipica del vostro modo di guardare le ragioni delle opposizioni, si svolge il voto su questo emendamento, credo che comunque qualcuno nel Paese stia ad ascoltare cosa avviene in quest'Aula e a decidere se alla fine ciò che qui avviene per volere della maggioranza e con il pieno consenso del Governo, su suggerimento del Governo - assai probabilmente, come qualcuno diceva a proposito dell'emendamento Fleres - davvero corrisponda agli interessi suoi propri o agli interessi della Nazione. Forse bisognerebbe stendere un velo pietoso sul fatto che nel testo originario dell'emendamento Fleres era addirittura previsto - udite! che tutti gli atti acquisiti in occasione della pratica per il rimpatrio dei capitali erano assolutamente inutilizzabili in ogni procedimento reale, per qualunque reato, in qualunque stato e grado si trovasse quel procedimento. Questa norma è saltata e immagino sia saltata di fronte ad un'opposizione molto netta da parte di chi controlla anche la costituzionalità dei testi che vengono emessi dal Governo e portati qui per l'approvazione. Ma quello che resta non è meglio, lasciatemelo dire!

attraverso i quali operava Sindona e per avere scoperto i quali, e la loro combinazione criminale e messa in opera, Ambrosoli fu ucciso. Stiamo parlando quindi di una materia che già solo in questo e solo per questo fa pensare al fatto che l'attuale Governo non ha nessuna memoria della storia del nostro Paese e ricade ogni volta negli stessi errori, non solo smentendo se stesso ma anche il fatto che questo Paese aveva detto: «Mai più può accadere, mai più dovrà accadere». E voi lo fate con la serenità, la superficialità e la insensatezza, lasciatemelo dire, che vi contraddistingue quando maneggiate questa materia. Voi, dunque, consentite di far rientrare i capitali dall'estero pagando soltanto il 5 per cento e facendo in modo che qualora si venisse a scoprire da queste operazioni che sono state violate norme molto gravi del nostro sistema, dai reati tributari a quelli molto gravi che vi hanno citato, questi non saranno punibili. Ma cosa sono le cause di non punibilità nel nostro sistema? Perché, ad un certo punto, il legislatore ha deciso che una determinata condotta criminale non deve essere perseguita? Andiamo a vedere. Alcune cause sono già elencate nel codice penale. Non è punibile, per esempio, chi non ha la capacità di intendere e di volere, oppure la moglie o il fratello che testimonia il falso rispetto allo stretto congiunto. Ma poi le altre cause di non punibilità quali sono? È vietato al legislatore di introdurne altre? No, non è vietato, però ogni volta il legislatore deve fare un contemperamento, un bilanciamento molto attento,

invece visto che ci stiamo infilando esattamente in quel nodo, per troppo tempo e per molti versi ancora oscuro, della storia italiana, caratterizzato da un intreccio tragico tra capitale, illecito, malaffare, mafia, poteri occulti.

e mi spiace ascoltare il ministro Tremonti quando parla della necessità di adottare il crisma della legalità nell'agire dell'economia:

la estemporanea, improvvisa e creativa fantasia del senatore Fleres che è stato messo al mondo. E poi ha anche ragione, lasciatemelo dire, il senatore D'Ambrosio: è una questione che era già stata sollevata nel 2002 quando faceste l'altro condono fiscale. In questo Paese si fa l'ira di Dio ogni volta che si discute dei temi della legalità e della sicurezza e voi, che l'indulto lo avete votato, ribaltate l'accusa da questa parte. Ovviamente, poi non andate neanche a guardarvi i dati, dai quali si evince che l'indulto ha abbattuto di due terzi la recidiva. Ma non è questo il problema: adoperate le armi della legalità e della sicurezza come una delle spine dorsali della vostra azione, ma questa porcheria che cosa è? È la negazione di ogni principio di legalità, e lo fate in disprezzo di ogni principio di equità! Ditelo agli italiani che togliete loro i soldi dalle tasche (come ogni Governo deve fare per finanziare la spesa pubblica, che non siete neanche in grado di governare) e che però a questi capitalisti, e ai tanti criminali che lì dentro si nascondono, a quelli che hanno levato capannoni, stabilimenti industriali, posti di lavoro e ricchezza ricchezza per il Paese, date un premio, non soltanto facendo loro pagare solo il 5 per cento, ma anche abbonando loro tutti i reati che possono avere commesso, perché, poverini, se no non si invogliano. E non riflettete anche su un'altra questione:

alcuni principi fondamentali di ogni convivenza civile, come quello di pagare le tasse, la solidarietà nazionale, il fatto che ciascuno produce per sé e per la propria famiglia ma anche per il proprio Paese, il fatto che l'impresa crea lavoro, l'esigenza che il denaro resti in questo Paese

da questo Governo per ogni azione che abbiano commesso! Allora, anche in ragione delle osservazioni che sono state fatte, poiché sul tema della legalità - da quando vi siete insediati e, prima ancora, in campagna elettorale - avete preteso

grande rilevanza della norma che ci accingiamo, o meglio, che la maggioranza si accinge ad approvare, chiediamo un pronunciamento, una valutazione, un parere della Commissione giustizia

alle categorie dell'indulto o dell'amnistia, riteniamo che sia necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione. Anche su questo punto vorremmo un suo chiaro pronunciamento.

Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte ad una norma abietta, che calpesta calpesta tutte le regole che uno Stato di diritto deve invece assolutamente rispettare favorisce il riciclaggio, un reato proprio delle organizzazioni criminali. Quindi, mi pare che il Ministro della giustizia, che ha tanto a cuore la battaglia - almeno così sostiene a parole - contro le organizzazioni criminali,

esonera dall'obbligo di denunzia delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio, di finanziamento al terrorismo, interne, internazionali e quant'altro,

si esprimono facendo riferimento ad una loro collegialità; non può essere supposta una diversa impostazione o valutazione e comunque non può essere fatto dal punto di vista delle procedure e dei Regolamenti. Per tali motivi, la Presidenza non può accedere alle richieste

Presidente, nessuno è contrario a momenti di concitazione, che in Aula ci possono essere. Ma l'insulto personale in quest'Aula non c'è. Ci sono stati degli atti e dei gesti in passato che hanno descritto le pagine più brutte dell'antiparlamentarismo; non le dobbiamo rinnovare per la distrazione della Presidenza. Nessuno vuole vedere in quest'Aula dei gesti, che vengono da dei senatori, senza che siano ripresi. Quindi prego la Presidenza di informarsi su quello che è successo e di esprimersi in proposito. Una cosa è la concitazione, altra cosa è l'insulto. la Presidenza, per quanto ha visto, quando il senatore Garaffa (se fa riferimento a lui) ha fatto dei gesti, lo ha richiamato ed è a verbale. Quando i senatori escono dall'Aula, non è che la Presidenza è distratta. C'è un gruppo di senatori che sta uscendo: la Presidenza non è distratta, ma non ha visto, che è una cosa diversa.

sono contrario, oggi, ieri e domani, a gesti di insulto che ledono la dignità del Senato. E siccome non credo che gesti negativi del passato facciano amnistia sul futuro, sono contrario anche ora e anche in futuro. Dopodiché, non avendo visto, se qualcuno informerà la Presidenza su quanto è avvenuto, la Presidenza valuterà e riferirà al presidente Schifani. Non ero distratto, ma non ho visto; sono due cose diverse.

fa riferimento ai poteri e alle competenze della procura presso la Corte dei conti e modifica in particolare i commi 30-*ter* e 34 dell'articolo 17 del cosiddetto decreto-legge anticrisi.

del primo testo che era stato proposto. Ricordo in Aula che già la Commissione giustizia aveva proposto all'epoca alcune modifiche e, in maniera peraltro molto garbata, anche il Servizio studi del Senato aveva sollevato perplessità sulle modifiche introdotte nell'ambito del nuovo decreto-legge. C'è stato e c'è ancora da parte nostra un richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare alla sentenza della Consulta del 2005 che viene interpretata scorrettamente e che viene piegata alle vostre esigenze. Continua, quindi, il vostro tentativo di paralizzare,

La Corte costituzionale in questa sentenza segnala in particolare che, nell'ambito dei poteri spettanti nei giudizi di responsabilità per danno erariale, l'ampio potere che il procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente - lo sottolineo perché così letteralmente dice la Consulta - configuranti illeciti produttivi di danno erariale. Dunque, la specificazione che voi imponete va contro questa interpretazione della Corte costituzionale. È un motivo in più di illegittimità costituzionale secondo l'interpretazione della Consulta che si vuole in questo momento intendersi nel senso che state continuando ad espropriare la Corte dei conti dei suoi costituzionali poteri di controllo. prosegue nel tentativo di gerarchizzazione della Corte dei conti, già parzialmente realizzato dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, la cosiddetta legge Brunetta, intervenuta in modo forte sulle competenze, sulla struttura e sulla e sulla composizione dell'organo di vertice della magistratura contabile, dando luogo ad una normativa contenente disposizioni in contraddizione tra loro, insufficienti e sicuramente non organiche. suddetta legge del 2009 ha modificato la coerenza del sistema costituzionale e di controllo esterno della Corte dei conti, che viene ad essere asservito e subordinato soprattutto al Governo centrale ma anche locale

la legge n. 15 del 2009, interviene di nuovo pesantemente sulle funzioni e sull'ordinamento della Corte, in contrasto con le esigenze e con le garanzie poste dalla Costituzione, nonché con i princìpi posti a presidio delle magistrature, in questo caso contabili, continuando ad introdurre princìpi e criteri gerarchici accentratori in modo non compatibile con i richiamati principi costituzionali. Per questi motivi, il Partito Democratico voterà a favore della soppressione

**Il Senato non approva.**

il mio voto su quell'emendamento era contrario.

definendo un percorso condiviso tra maggioranza ed opposizione. L'aver introdotto per via parlamentare uno stravolgimento di norme estremamente importanti che riguardano il rimpatrio e la regolarizzazione di capitali illecitamente trasferiti all'estero, senza che su questo vi sia stata la possibilità di un confronto di merito, attraverso un emendamento proposto surrettiziamente all'ultimo minuto per consentire una sorta di indulto mascherato (cancellando peraltro quelle norme del pacchetto sicurezza che insieme abbiamo costruito per migliorare la qualità e quantità del contrasto al crimine organizzato, con particolare riferimento all'aggressione ai patrimoni mafiosi e al riciclaggio del denaro al riciclaggio del denaro illecitamente prodotto dalle organizzazioni criminali), ha seriamente compromesso non solo la dinamica dei rapporti parlamentari, ma anche il merito di questo provvedimento che ovviamente non possiamo e non intendiamo votare.

con quanto quotidianamente e giustamente il Ministro dell'interno dichiara in materia di contrasto alla criminalità organizzata, con quanto giustamente e legittimamente il Ministro della giustizia afferma in materia di contrasto e di aggressione ai patrimoni mafiosi, con quanto

intercettazione dei flussi di capitale - e sono tanti anche nel nostro Paese - funzionali al finanziamento del terrorismo internazionale.

attraverso cui si finanzia il terrorismo islamico nel nostro Paese; quando consentite con leggerezza l'approvazione di tali norme senza valutarne l'impatto, noi, che anche sul tema dello scudo ci siamo pronunciati in linea di principio a favore, ci troviamo disgustati a dover votare contro, e ci dispiace che voi non siate altrettanto disgustati.

e, a nostro giudizio, devastanti che esso produrrà. Dobbiamo innanzitutto fare chiarezza su quanto si sta facendo questa mattina, con un semplice dato, oggettivo, inconfutabile ed immune da qualsiasi faziosità. Siamo all'ottavo decreto-legge anticrisi, partendo dall'estate scorsa, in piena crisi internazionale, da una finanziaria anticipata e presentata, con una retorica alla quale ormai siamo avvezzi, come un moderno ed efficiente strumento della sessione di bilancio, per arrivare ora a una finanziaria superleggera, *light*, *soft*, che in italiano significa pochi articoli, ma anche niente soldi. Nel mezzo abbiamo avuto, in tutti questi mesi, una manovra finanziaria permanente ed inconcludente, fatta di norme vuote, di risposte truccate, di scelte pilotate scientificamente a difesa degli interessi di pochi e a danno di molti;

e che non sa tenere conto, fatto ancora più grave, che le Regioni hanno disertato l'altro ieri l'incontro con il Governo considerandolo ormai inutile.

vengono concessi dalla Commissione europea solo se abbinati a politiche attive del lavoro; ciò significa che le Regioni, per ottemperare alle disposizioni di Bruxelles, devono attivarsi con corsi di formazione quanto meno di dubbia efficacia. Stiamo parlando di una manovra finanziaria che, nonostante i Tremonti *bond*, non sa tener conto che nei primi sei mesi dell'anno all'interno dell'area euro un'impresa su dieci si è vista respingere una richiesta di finanziamento; che circa un terzo delle piccole imprese ha denunciato un peggioramento delle condizioni di accesso al credito (l'Italia assieme alla Spagna è il Paese con la quota più consistente). Questa criticità non è denunciata da un gruppo eversivo o di opposizione, ma dalla Banca centrale europea. Allora, di fronte alla necessità di misure fiscali forti a favore dei redditi dei lavoratori e dei pensionati, di un alleggerimento dell'IRPEF per queste categorie, di un raddoppio della durata della cassa integrazione, di una riforma degli ammortizzatori sociali, di un'estensione alle famiglie della moratoria sui debiti concessa alle imprese, di un alleggerimento del patto di stabilità dei Comuni virtuosi e di fronte alle Regioni che stanno chiedendo la restituzione dei Fondi aree sottoutilizzate (FAS) per avere più risorse per la sanità e per fronteggiare i tagli alla scuola, il Governo conferma - lo ha fatto con questo decreto e lo farà con la prossima manovra - una politica economica che il ministro Tremonti ha definito prudente.

I soldi ci sono o ci mancano? Mi limito a rispondere alla seconda domanda, e mi rivolgo ai colleghi dell'opposizione e della maggioranza: è sorprendente il rapporto 2009 della Ragioneria dello Stato sulla spesa delle amministrazioni centrali, dal quale emerge che l'anno scorso nelle casse dei Ministeri sono rimasti 90 miliardi di euro di residui non utilizzati, di cui il 20 per cento è formato da risorse mantenute in bilancio per l'esercizio successivo.

Nel campo dell'energia manca una seria programmazione; si discute di carbone, di rigassificatori e di biomasse, senza che nessuno stabilisca il quanto e il dove e senza un piano energetico nazionale di riferimento. Le modifiche normative più radicali sono state camuffate, anche in questo decreto, da una veste di decisionismo, di semplificazione, di generico adeguamento a parametri europei, senza rendersi conto che l'Italia ha perso sul piano legislativo il concetto di ambiente come valore costituzionalmente garantito. È chiaro il timore che il Governo possa decidere tutto da solo, limitandosi a chiedere agli enti locali un parere non vincolante. Ne sanno qualcosa

che con gli articoli 25 e 26 dà di fatto mano libera al Governo per la localizzazione di nuove centrali nucleari. Per quanto riguarda lo scudo fiscale - lettera *b)* dell'articolo 1, la definizione di riciclaggio di Stato fatta dall'autorevolezza, dalla competenza e dalla capacità del senatore Lannutti non rende a sufficienza l'idea di quanto si sta facendo. Si tratta in realtà di un furto ai danni dello Stato, anzi di un doppio furto! Quanto costa far rientrare i capitali all'estero? Per ogni 100 euro detenuti all'estero, in Italia il costo sarà di 5 euro

del senatore Fleres - è quello di rendere il più possibile appetibile la sanatoria per il rientro dei capitali, allettando i disonesti. Bisogna chiamare le cose con il loro vero nome. Nei reati tributari che sono scudati non rientrano soltanto la dichiarazione infedele o l'omessa dichiarazione, ma anche la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o documenti di operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, falsità in registri, false comunicazioni in danno alle società, dei soci e dei creditori, l'occultamento e la distruzione di documenti contabili.

Il risultato finale è che si incoraggia l'evasione fiscale, perché se i disonesti riescono a tornare nella legalità pagando una piccola quota di quanto avrebbero dovuto, si crea inevitabilmente un clima lassista, permissivo e un'aspettativa di altri condoni che fa perdere allo Stato più risorse di quanto nell'immediato spera di incassare. Questa non è la denuncia di un Gruppo consiliare radicale, eversivo o fazioso. Questo è l'allarme lanciato dalla Corte dei conti davanti alle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato sin dal mese di luglio, quando ha dichiarato a chiare lettere che lo scudo fiscale può essere percepito dai contribuenti come un segnale di attenuazione del rigore fiscale e addirittura una promessa di nuovi condoni, al punto che gli effetti della deterrenza delle misure antievasione rischierebbero di essere largamente vanificati in un momento in cui la lotta all'evasione deve trasformarsi in uno strumento di bilancio. decreto-legge, sulla Corte dei conti. Qui, signor Presidente, si attua il paradosso dei paradossi: limitando l'azione della magistratura contabile, che può iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale solo a fronte di una specifica e concreta notizia di danno, si introducono delle disposizioni assurde con conseguenze perverse. In un decreto‑legge che si definisce anticrisi e che dovrebbe, tra l'altro, aiutare a recuperare soldi, la stretta sulla Corte dei conti in realtà li farà perdere. inchieste su dieci saranno paralizzate già dalla fase di apertura. A nulla, quindi, è servito l'invito del presidente Napolitano. Questo è quanto. Il Parlamento, signor Presidente, ha quindi il dovere di far aprire gli occhi al Governo; è un dovere tanto più necessario e urgente perché nel nostro Paese l'emergenza lavoro e l'aumento della disoccupazione devono ancora venire. La cosa più drammatica non sono i dati, che ci fornisce l'OCSE, di un milione di disoccupati in più, ma il fatto che l'impatto della crisi sul mercato del lavoro italiano è stato fino ad oggi moderato rispetto agli altri Paesi solo perché un gran numero di persone, soprattutto del Sud, ha perso la speranza e ha rinunciato a cercare lavoro. Questo è il dramma con il quale questo Parlamento deve confrontarsi! Il Parlamento poi può anche rassicurare il Governo. Abbiamo letto in questi giorni sulla stampa che alcuni autorevoli esponenti del Governo temono da parte dell'opposizione un colpo di Stato. Chi come noi visita i territori e viene a contatto con i cittadini assicura a questo Parlamento che gli italiani in questo momento non sono preoccupati degli effetti devastanti di un colpo di Stato, sono molto più preoccupati - questo decreto ne è la prova - degli effetti devastanti dei colpi di sole di chi dovrebbe avere la responsabilità delle scelte. Signor Presidente, colleghi senatori, gentili membri del Governo, il Gruppo Lega Nord-Padania voterà a favore delle disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi. Quanto ci apprestiamo a votare oggi - ricordo le modifiche all'articolo 4 in materia di interventi urgenti per le reti e l'energia e in materia di impatto delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato e le modifiche all'articolo 17 in materia di disciplina della Corte dei conti - non può essere assolutamente valutate in modo disgiunto dal provvedimento approvato in quest'Aula lo scorso 1° agosto. sono state le polemiche in queste settimane sulle modalità di approvazione di quelle norme, sulle quali il Governo ha prima posto la fiducia e poi emanato subito dopo un decreto‑legge correttivo. Non mi fermerei all'aspetto estetico ma guarderei soprattutto alla sostanza. Vorrei sottolineare come il Governo e la Lega Nord in questo momento godano della fiducia di chi vive in questo Paese, in particolare del sistema produttivo, per il quale stiamo portando avanti, e non da oggi, una politica di sostegno al sistema delle imprese, ma anche equità e rigore nei conti pubblici e defiscalizzazione. del tutto contraria a quella dell'opposizione, che invece continua a proporre l'aumento del deficit e l'imposizione fiscale. Abbiamo affrontato con un insieme di misure strutturali e congiunturali la più grave crisi economica del dopoguerra. Non dobbiamo dimenticarcelo. Ricordiamo la manovra di sostegno del sistema finanziario, volta a immettere liquidità nel sistema bancario, quando la crisi ha trasmesso i suoi effetti sull'economia reale, è arrivato un provvedimento anticiclico, che ha incentivato l'acquisto di automobili, ha potenziato la cassa integrazione ed ha rimodulato le imposte gravanti sulle imprese. Non voglio dilungarmi qua in una lunga lista, ma vorrei solo ricordare come il provvedimento anticrisi abbia lavorato sulla lotta agli sprechi nella pubblica amministrazione, per il sostegno alle imprese attraverso la detassazione degli investimenti in macchinari, il sostegno alla capitalizzazione e disposizioni sull'anticipazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa. Questo per ricordarne soltanto alcuni. Per quanto riguarda il tema del lavoro, penso siano siano assolutamente evidenti i benefici effetti della politica adottata a sostegno della cassa integrazione. Vanno, inoltre, considerate positivamente le misure che premiano le imprese che non licenziano, il sostegno alle iniziative imprenditoriali di coloro che perdono il posto di lavoro. Riteniamo che uno degli effetti importanti queste misure anticrisi sia soprattutto che si è operato sui due versanti: sulla domanda e sull'offerta. Meritano di essere menzionati l'intervento per la patrimonializzazione delle imprese, la riforma previdenziale, la

dei colleghi del centrosinistra, che hanno determinato le condizioni perché gli imprenditori andassero a cercare delle alternative. Ritengo che ciò possa non essere giusto né eticamente corretto. Però questo è successo. Che cosa si fa adesso? Bisogna cercare di invertire la tendenza. Quindi, dalla fuga dei capitali

è vero che andiamo ad attuare delle norme che possono essere magari considerate moralmente poco corrette, ma oggi pensiamo a quello che è stato il motivo per cui questi capitali sono andati all'estero, ed oggi il nostro dovere è fare in modo che questi capitali rientrino per essere la base della ripresa di questo Paese. Abbiamo bisogno di capitali, di persone e di imprenditori che investono ed abbiano fiducia in questo Stato. Quel che si sta cercando di fare con questo provvedimento ritengo vada in questa direzione. Sul merito di queste misure correttive, come Lega Nord, siamo soddisfatti che il Governo abbia recepito alcune nostre proposte riguardanti per esempio l'incentivazione del trasporto fluviale del GPL. Altro aspetto che riteniamo molto importante, e che ha trovato condivisione dei colleghi, non solo in Commissione ma anche in Aula, è chiarire alcuni aspetti legati all'errata applicazione dell'articolo 17, comma 30 della legge di conversione da parte di alcune di alcune amministrazioni locali, che ritenendo di rientrare nell'ambito applicativo di questa disposizione stanno trasmettendo provvedimenti di attribuzione di incarichi per il controllo preventivo di legittimità alla sezione di controllo della Corte dei conti; ciò in contraddizione con l'abolizione di qualsiasi forma di controllo preventivo degli atti degli enti locali, stabilita dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Mi avvio rapidamente alla conclusione di questo mio breve intervento sottolineando con forza come alle manovre economiche varate dal Governo, con il fattivo contributo della Lega Nord, vadano aggiunte le riforme istituzionali in materia di federalismo, di contabilità pubblica e di codice delle autonomie. grazie al nostro importante contributo, il Governo e la maggioranza stanno dunque continuando con determinazione nel processo di costruzione di uno Stato più snello, più efficiente, equo e federale*.

di gravi conflitti insorti all'interno del Governo su diverse misure, *in primis* quelle relative alle norme sui poteri autorizzatori delle reti dell'energia, e soprattutto dei rilievi di incostituzionalità, informalmente ma tempestivamente e correttamente espressi dalla Presidenza della Repubblica, il Governo e la sua maggioranza, piuttosto che rimediare con la lettura che a fine luglio era in corso al Senato, decisero di intervenire con un successivo decreto correttivo, quello appunto che oggi stiamo esaminando. Una grave forzatura costituzionale che si sostanziava in una vera e propria terza lettura operata dal Governo al solo scopo di non turbare il programma feriale della Camera dei deputati. Il Senato, ancora una volta, veniva chiamato a ratificare con il voto di fiducia un testo blindato che poteva essere agevolmente emendato con qualche giorno in più di lavoro parlamentare. Invocando un unico, anche se alquanto diverso e circoscritto, precedente, fu varato questo decreto, che accoglieva la modifica delle più macroscopiche anomalie contenute nella legge n. del 2009. Ritenevamo, e in tal senso ci siamo espressi nelle Commissioni riunite 5a e 6a, che l'intervento correttivo avrebbe richiesto modificazioni più incisive,

le norme sulla procedura di accertamento della responsabilità contabile dei pubblici amministratori, fortemente limitata dalle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati. Erano e sono rimaste immodificate le norme che introducono una sorta di sbarramento all'ingresso nell'esercizio dell'azione contabile avanti alle procure della Corte dei conti, prescrivendo la necessità di una notizia di danno specifica e precisa quale condizione di procedibilità. Uno sbarramento che inciderà su decine dì migliaia di procedimenti pendenti, essendo stata introdotta *ex post* la sanzione di nullità per gli atti istruttori e processuali sin qui compiuti a seguito di notizie di danno prive dell'iniziale carattere di specificità e precisione.

con la conseguenza che le sezioni regionali della Corte dei conti passeranno i prossimi mesi e anni a parare i colpi delle difese sulle eccezioni di nullità e a stabilire se la notizia di danno è concreta o non è concreta, e ciò prima di avviare le attività di indagine. Con il risultato finale di una fortissima limitazione del deterrente più incisivo all'uso distorto dei poteri pubblici, quello appunto della responsabilità contabile. Sull'aspetto più controverso del provvedimento, quello dello scudo fiscale e dei connessi aspetti condonistici e penali è stato detto tutto ciò che c'èra da dire dalla presidente Finocchiaro e dagli altri colleghi che sono intervenuti. Mi limito a segnalare l'evoluzione del pensiero della maggioranza e del Governo. A fronte della certa incidenza della disposizione sull'inutilizzabilità dello scudo nei procedimenti anche penali e dei conseguenti profili di incostituzionalità autorevolmente rilevati, il Governo era intervenuto con l'unica modifica possibile, quella cioè dell'espressa esclusione dei procedimenti in corso. Con una successione di testi emendativi esaminati dalle Commissioni di merito, la maggioranza, con l'espressa adesione del Governo, aveva dapprima addirittura esteso il beneficio dell'inutilizzabilità dello scudo a tutti i procedimenti penali, tentativo che è stato vanificato a seguito della nostra ferma opposizione nelle Commissioni la scorsa settimana, e successivamente è venuta assestandosi sulla norma oggi approvata in Aula. Non si può prevedere l'inutilizzabilità dello scudo nei processi penali pendenti? Questo era il quesito e questa era la norma correttiva contenuta nel testo originario del decreto. Allora eliminiamo i processi penali con un'estesa depenalizzazione di un numero consistente di reati, anche gravi, strumentali all'illecita esportazione di capitali all'estero e all'evasione delle imposte. Tutti i proclami del Ministro dell'economia nei mesi scorsi in base ai quali tutto sarebbe stato concordato in sede Ecofin e non sarebbero state percorse vecchie strade sul rientro dei capitali sono stati platealmente contraddetti. Il Presidente del Consiglio dichiarò a Bruxelles, il 20 marzo scorso, al termine del vertice dell'Unione Europea, che «l'Italia prenderà in considerazione l'ipotesi di ricorrere ad un nuovo scudo fiscale solo se la misura verrà messa in campo dall'Europa» e aggiungeva che «la misura non dovrà essere una semplice riedizione dei vecchi scudi del 2001 Il 12 luglio scorso, il quotidiano «la Repubblica» pubblicò un articolo sullo scudo fiscale, sostenendo che vi era un piano del Governo per varare uno scudo contenente il condono per il falso in bilancio. bilancio. Il ministro Tremonti il giorno stesso rispose testualmente: «L'articolo pubblicato da "la Repubblica" è totalmente falso». Ora è facile constatare che chi ha dichiarato pubblicamente il falso sono stati il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia. Per una casualità, la norma è stata approvata nel giorno stesso del varo della legge finanziaria, ieri, in Consiglio una manovra vuota che registra il più grande peggioramento dei conti pubblici dal 1992 ad oggi. Neanche gli impegni finanziari minimali risultano rispettati con il testo approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che ci è stato anticipato dalle dichiarazioni del ministro Tremonti e del Presidente del Consiglio. Occorrono proroghe di incentivi vari vigenti da anni o di quelli più recentemente introdotti? Occorrono le risorse per i contratti del pubblico impiego? Ci penseremo successivamente, magari con il decreto milleproroghe: questo ha dichiarato il Ministro dell'economia. E degli ulteriori fondi promessi per il terremoto in Abruzzo neanche l'ombra nella legge finanziaria, né in altri provvedimenti. La verità è quindi chiara: la politica economica e di bilancio del Governo e - certo - anche la crisi stanno portando il bilancio pubblico ad un passo dalla bancarotta. Non si spiega altrimenti l'utilizzo dei 525 milioni di euro che i terremotati abruzzesi dovrebbero, con larghissimo anticipo, riversare alle casse dello Stato per finanziare le misure anticrisi. Una vergogna senza precedenti, aggravata dal fatto che la promessa di modifica della norma è rimasta a tutt'oggi inattuata, fino al voto contrario di oggi su un nostro specifico emendamento sul punto. Le sole risorse disponibili saranno quindi quelle che i furbi, con un robusto premio, metteranno - se ciò avverrà - a disposizione dello Stato. Così si spiega l'anticipo della scadenza al 15 dicembre e l'indulto agli evasori e ai falsificatori di bilanci e fatture. Questa è la verità, signori del Governo e della maggioranza! Il combinato disposto delle misure del decreto corretto e di quello correttivo connotano la politica economica del Governo più di molte chiacchiere e proclami. Il Parlamento è svilito, la Costituzione viene continuamente forzata, la politica economica del Governo ripercorre vecchie strade, cioè i condoni per tappare i buchi del bilancio pubblico.

il Gruppo del Popolo della Libertà voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. Voterà a favore, perché ha rispetto del ruolo del Parlamento; voterà a favore, perché è consapevole del fatto che il nostro sistema normativo è assai complesso e, dunque, non è difficile che si verifichi, come in questo caso, la necessità di correggere disposizioni già varate, sia pure nel recente passato. È accaduto ai precedenti Governi e, pertanto, non credo ci si possa meravigliare di un passaggio di questo genere. Il Gruppo voterà sì, perché ha ritenuto giusto ascoltare chi auspicava una più ampia assunzione di responsabilità nelle decisioni riguardanti gli interventi urgenti relativi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia elettrica. Voterà sì, perché è convinto che sia compito del Parlamento evitare equivoci interpretativi circa la vicenda del ponte sullo Stretto di Messina; anche perché; signor Presidente, noi vogliamo fare il ponte e lo vogliamo fare perché crediamo nella capacità che quest'opera ha circa il rilancio delle attività economiche ed il miglioramento della mobilità stradale e ferroviaria nel Mezzogiorno ed in Sicilia. Voterà sì, perché si è reso conto che le norme, recentemente votate in materia di esercizio dell'azione di danno erariale, potevano dare adito ad equivoci interpretativi: dunque era ed è giusto correggerle. Voterà sì, perché non vuole che esistano coni d'ombra nell'azione di controllo preventivo della Corte dei conti e nel trasparente rapporto tra controllore e controllato. Voterà sì, perché cambiare idea, tenere conto delle idee degli altri, correggere le proprie opinioni, alla luce delle esperienze maturate, individuare soluzioni adeguate rispetto a problemi emergenti sono segni di intelligenza e soprattutto di realismo ed oggettività. La nostra azione politica non è certo caratterizzata né da rigorosi ideologismi, né da anacronistici fideismi, né da pericolose ipocrisie o indifendibili bigottismi istituzionali. Se vogliamo essere moderni, se vogliamo affrontare i problemi complessi del Paese, se vogliamo contribuire ad uscire dalla crisi economica, dopo essere riusciti a contenerne i danni con i provvedimenti adottati a tutela dei più deboli da parte del Governo (dobbiamo tutti ricordare l'Esecutivo ha affrontato di petto la crisi e ha evitato che essa degenerasse creando problemi al Paese), abbiamo bisogno di bandire dai nostri processi mentali il concetto di ipocrisia. L'ipocrisia è l'agonia dei valori, di qualsiasi valore; essa verrebbe pagata dai cittadini di quello Stato che dovesse fingere di ignorare i problemi reali. Signor Presidente, illustri componenti del Governo, onorevoli senatori, proprio perché, da tempo, abbiamo segnalato i pericoli dell'ipocrisia applicata alla politica e poiché abbiamo il dovere di ascoltare le opinioni delle alte cariche dello Stato, pur contestualizzandone il contenuto, voteremo sì anche per le novità introdotte in materia di scudo fiscale. Il provvedimento dei mesi scorsi aveva bisogno di fare un tagliando; il Presidente della Repubblica ha segnalato l'opportunità di apportare qualche correzione alle disposizioni presentate nel luglio scorso, ed era giusto tenerne conto. Era necessario raccogliere l'invito delle autorità internazionali circa le azioni di contrasto ai reati finanziari e al fenomeno di esportazione di valuta. La nostra economia ha bisogno di poter godere di capitali rientrati dall'estero che altrimenti, onorevoli colleghi dell'opposizione, non produrrebbero alcunché, se non stucchevoli polemiche come quelle udite oggi. Le finanze pubbliche possono fruire delle somme connesse con il rientro di questi capitali, magari per investirle nello sviluppo del Paese. Certe nostre imprese devono poter recuperare la via della legalità e devono poterla mantenere per sempre. Gli accordi internazionali devono poter ridurre il fenomeno dei paradisi fiscali. Questi sono alcuni degli ingredienti di un ragionamento che aveva bisogno di essere fatto fino in fondo e non per titoli, né per *slogan*, abbiamo bisogno di comprendere le dinamiche dello Stato e ciò che ha provocato la fuga di capitali, a cominciare dalla ben nota tendenza a tassare e tartassare, messa in piedi dai precedenti Governi di sinistra. Questa non è certo una giustificazione per chi comunque ha eluso la legge, ma è una constatazione. Così come è una constatazione che questi capitali sono emigrati a causa della sfiducia dell'imprenditoria, provocata dai provvedimenti del centrosinistra, e che, se non rientrano, restano dove oggi si trovano e continuano a non produrre nulla per il fisco italiano. onorevoli colleghi, si chiede perché bisogna sconfiggere l'ipocrisia, questo è un esempio. Bisogna essere realisti e, magari, contenere giudizi affrettati affrettati di pessimo gusto, come quelli di qualche guitto che ho visto esibirsi in Aula questa mattina. Ecco perché bisogna sconfiggere l'ipocrisia. L'ipocrisia è quella di chi tocca il fuoco con le mani degli altri e poi dice che c'è il rischio di ustioni. Vedete, colleghi, se si vuole ripulire il Paese, ci vuole qualcuno che faccia il netturbino. Non è il netturbino che ha sporcato il Paese, non è sua la responsabilità, di chi ha prodotto i rifiuti. La responsabilità è di chi quei rifiuti li ha prodotti, di chi li ha provocati, di chi ne ha favorito l'accumulo; non certo di chi deve intervenire per far sì che quei rifiuti non producano altri effetti. Quello che voteremo è un provvedimento straordinario, è un provvedimento scomodo, ma necessario. Lo facciamo perché il nostro non è un comportamento ipocrita, il nostro è un comportamento realistico, in linea con quello che sta accadendo sul piano internazionale, sia in questa materia, sia rispetto alle prospettive di cui si è parlato nel corso del dibattito. Su questi temi serve ripartire da zero, evitando che il fenomeno si ripeta. Ci auguriamo che questo azzeramento ci sia, ci auguriamo che i capitali rientrino, che le somme vengano investite nella nostra economia e che questo - per così dire - "sacrificio politico" (perché tale è un provvedimento di questo tipo) raggiunga i risultati auspicati. Dunque (e concludo, onorevoli senatori), voteremo sì contro il mantenimento di tanti e inutili equivoci; voteremo sì contro le ridicole strumentalizzazioni; voteremo sì contro la retorica da piazza, ma anche contro la retorica da salotto, che forse è la peggiore. voteremo sì contro l'ipocrisia di chi non ha nessuna idea di responsabilità e di governo, non pone soluzioni alternative, forse userà pure lo scudo e pretende persino di dare lezioni agli altri.

Desidero ricordare a tutti colleghi che, in conformità con quanto deliberato dal Comitato per la sicurezza, in adempimento del mandato ricevuto dal Consiglio di Presidenza, il prossimo 30 settembre cesserà la validità dei permessi di accesso concessi ai collaboratori dei senatori sulla base della precedente normativa. Da tale data, di conseguenza, tutti i collaboratori che non avranno ottenuto il rilascio del nuovo *badge*, a seguito della consegna della documentazione prevista dalla delibera del Comitato per la sicurezza del 27 maggio 2009, potranno accedere ai palazzi soltanto come ospiti, sulla base di accrediti giornalieri, e perderanno la possibilità di fruire dei servizi di mensa e degli accessi alla rete informatica. Ricordo che al momento sono assai pochi i colleghi che hanno provveduto a quanto sopra ricordato.

L'emendamento del quale si è molto discusso, ossia l'emendamento 1.3500, consente la deroga all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il decreto legislativo in questione non è altro che l'attuazione della direttiva della Comunità europea concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70 della Comunità europea che ne reca misure di esecuzione. Abbiamo introdotto una deroga ed una possibilità di violazione

dando luogo alla possibilità di creazione di fondi destinati ad attività terroristica che possono mettere in pericolo

mi rifiuto di partecipare al voto, come espressione di estrema protesta rispetto ad un provvedimento che, oltre a non avere un connotato etico, offende la sicurezza del nostro Paese e manifesta integralmente la sua anti-italianità.

dei campi ormeggio da parte degli enti preposti sulla base delle prescrizioni dell'Istituto idrografico della Marina, esso prende in considerazione anche la posizione e le caratteristiche dei campi, che devono essere comunicate dagli

il Gruppo dell'Italia dei Valori, nel corso dell'esame del provvedimento che oggi si vota, ha posto l'accento sulla necessità di coordinamento normativo, operativo e gestionale dei campi ormeggi attrezzati, al fine di evitare che i Comuni e le aree protette si avvalgano della facoltà concessa dalla presente legge in modo disomogeneo sul territorio nazionale e, soprattutto, in modo contraddittorio con gli obiettivi di tutela ambientale che ne sono alla base, non potendosi ragionevolmente passare da un regime di totale inaccessibilità ad una gestione caotica o frammentaria della pressione turistica e diportistica su aree sensibili. Miglioramenti su questo fronte sono oggettivamente intervenuti con l'approvazione di alcuni emendamenti ed ordini del giorno, pertanto faremo particolare attenzione alle modalità con cui la legge, una volta approvata, verrà applicata nei casi concreti. Restano nel complesso alcune incertezze sugli effetti che le disposizioni in esame potrebbero produrre sul demanio marittimo: alla luce dell'emendamento proposto dal relatore sulla invarianza dei costi per la finanza pubblica, ci sembra evidente che la gestione del regime concessorio, e cioè la scelta della gratuità od onerosità (poiché tutto il provvedimento è imperniato sulla libertà di scelta degli enti) dovrà essere particolarmente attenta. Nel complesso, esprimiamo un voto favorevole sul provvedimento in esame alla luce dei miglioramenti apportati in Commissione e in Aula, apprezzando anzitutto il fatto che finalmente sia approdato in Aula un provvedimento di iniziativa parlamentare e, per di più, dell'opposizione. Onorevoli Senatori, signor Presidente, il disegno di legge che abbiamo appena esaminato interviene sulla tutela dell'ambiente marino, che rappresenta per il nostro Paese un patrimonio inestimabile di risorse ambientali ed economiche. Lo sviluppo turistico delle nostre coste è strettamente legato sia con la qualità dell'ambiente marino sia con i servizi offerti alle attività turistiche. L'istituzione delle aree marine protette ha avuto infatti lo scopo di assicurare una tutela adeguata ed efficace degli ecosistemi marini e costieri, costantemente minacciati dalle attività antropiche, contrastando la riduzione delle risorse ittiche, assicurando il mantenimento e la conservazione della biodiversità e garantendo la protezione del territorio, senza però escludere le attività umane da tali aree. D'altra parte le aree protette, oltre ad essere quelle maggiormente sensibili e delicate, sono anche quelle maggiormente frequentate dai turisti, perché costituiscono veri poli di attrazione per la notevole varietà delle specie animali e vegetali e per le molteplici testimonianze storiche e paesaggistiche. L'eccessiva pressione turistica in questi tratti di costa, specialmente nel periodo estivo, ed in particolare l'ancoraggio selvaggio delle barche sui fondali, minacciano gli equilibri dell'ecosistema marino, arrecando danni irreparabili e disturbi che non consentono la rigenerazione delle risorse. Inoltre, la maggior parte delle aree marine protette e quelle intorno alle isole minori, per lo più situate nel Centro-Sud, soffre di una cronica carenza di infrastrutture da diporto e di approdi attrezzati o di porti turistici, fatto, questo, che pregiudica una corretta gestione delle coste e dei posti barca. In questo contesto si inserisce il disegno di legge approvato dalla Commissione ambiente, che, in alternativa o in aggiunta alle infrastrutture da diporto, permette di dotare le coste italiane di campi di ormeggio regolamentati *off shore*, a servizio della nautica da diporto, prevedendo un regime agevolato, ad esenzione concessoria. La proposta riprende analoghe iniziative sperimentate con successo in altre parti del Mediterraneo, ove sono avvertite analoghe esigenze. La Commissione ambiente ha svolto un proficuo lavoro in sede referente, convinta dell'importanza del disegno di legge che potrà incidere positivamente anche sulle disponibilità economiche degli enti gestori delle aree protette, in quanto destina i proventi, oltre che al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi di ormeggio, ad interventi che incrementano la protezione ambientale

a quanto avviene per le aree marine protette, possono istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione antropica. In questo modo, il disegno di legge riguarda tutto il territorio nazionale e non solo le aree marine protette e quelle di reperimento. La Lega Nord condivide gli obiettivi di tutela delle coste promossi dal presente disegno di legge e vota a favore del provvedimento.

dal lavoro di colleghi di altri Gruppi (in particolare, voglio ringraziare il presidente D'Alì e il senatore Alicata per il contributo importante che hanno dato per rendere spedito e rapido

Per molto, per troppo tempo, e in Italia forse più a lungo e con più inerzia che altrove, è prevalsa l'idea che difesa dell'ambiente e ragioni dello sviluppo fossero istanze tra loro in contrasto, e che di volta in volta chi fa le leggi, chi governa, chi amministra dovesse scegliere di privilegiare l'una o le altre. Con sempre maggiore evidenza si va invece dimostrando che così non è perché il degrado dell'ambiente rappresenta un costo, un disvalore anche in termini economici, e perché molto spesso le politiche, le scelte che rafforzano la tutela ambientale possono dare ottimi frutti anche sul terreno dello sviluppo economico duraturo e sostenibile. Un caso tipico di questo possibile circolo virtuoso è rappresentato proprio dal disegno di legge che ci accingiamo, mi auguro, ad approvare. Promuovere la realizzazione di campi ormeggio senza ancoraggio sui fondali nelle aree marine protette e in generale lungo i tratti più belli e delicati delle nostre coste consente infatti, ad un tempo, di tutelare meglio gli ecosistemi e la biodiversità del mare e delle coste italiani e di facilitare la fruizione turistica sostenibile di queste aree. Oggi in Italia vi sono più di 20 aree protette marine già istituite, che tutelano 200.000 ettari di mare e oltre 500 chilometri di costa. Se ad esse si aggiungono le aree già previste da leggi in vigore ma non ancora istituite, si arriva ad una percentuale di territorio costiero protetto superiore al 10 per cento dell'intera linea di costa nazionale. Forse l'habitat più caratteristico e prezioso che accomuna gran parte di questi ambienti è quello delle praterie di posidonia. La posidonia oceanica è probabilmente la singola specie più importante della fascia costiera del Mediterraneo: un solo metro quadrato di posidonieto produce 14 litri di ossigeno al giorno, e nelle praterie trovano rifugio, nutrimento e si riproducono oltre 1.200 specie animali e vegetali. Indicate dalla "direttiva habitat" del 1992 come uno degli ecosistemi a protezione prioritaria, le praterie di posidonia sono quasi ovunque in regressione a causa di impatti antropici di varia origine: inquinamento, pesca, urbanizzazione costiera e, per l'appunto, ancoraggi delle imbarcazioni. Incentivare, come fa questo disegno di legge, la sostituzione dell'ancoraggio sui fondali con l'ormeggio ai campi boa potrà aiutare a difendere di più e meglio le posidonie e, con esse, la qualità ambientale e paesaggistica e, spesso, l'unicità dei tratti meglio conservati del nostro ambiente costiero. Questo - ritorno al punto da cui sono partito, perché mi sta molto a cuore - è un grande, irrinunciabile interesse ambientale, ma è anche un interesse economico rilevante per il nostro Paese e una necessità vitale per il benessere delle comunità locali che vivono in queste aree costiere. Tanti esempi, sia positivi che negativi, dimostrano che difendere l'ambiente, proteggere e tutelare le bellezze naturali di cui l'Italia è così ricca, sono una condizione essenziale per dare un presente e un futuro solido all'economia turistica turistica e che, invece, disinteressarsi della qualità ambientale dei nostri territori, magari esponendoli a un'eccessiva pressione turistica o a una cementificazione senza limiti, inevitabilmente li svaluta anche sul piano turistico e, dunque, economico. Il mio Gruppo voterà, dunque, a favore di questo disegno di legge e io mi auguro che i principi che lo ispirano possano presto allargarsi rapidamente anche ad altri campi della legislazione e delle politiche ambientali. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del PdL desidero sottolineare alcuni aspetti, così come ha fatto anche il collega Della Seta, ed esprimere

che ne ha seguito l'*iter* con assoluta puntualità e che ha dato anche utili suggerimenti perché la proposta normativa trovasse una giusta collocazione nel quadro complessivo delle norme che riguardano tanto il demanio marittimo quanto le aree protette. Voglio sottolineare il dato politico da un punto di vista operativo. Finalmente andiamo a costruire un primo piccolo tassello di una normativa che vuole coniugare in maniera positiva e razionale, senza senza accedere ad alcun estremismo, l'aspetto della salvaguardia ambientale con quello dello sviluppo turistico, soprattutto delle zone

una delle voci importanti che, anche in un periodo come questo, reggono alle sfide della crisi economica e portano nei nostri territori ricchezze sempre più consistenti. Un modello di Un modello di approccio a queste tematiche che la Commissione si ripromette di seguire anche su temi altrettanto importanti quali quelli della disciplina della disciplina normativa specifica per le isole minori o della revisione della stessa normativa sugli enti parco e sulle aree marine protette che presto metteremo in cantiere. Vi è anche un altro un altro indirizzo che la Commissione vuole perseguire (mi riferisco alla Commissione perché ho sempre l'occasione di raccogliere le opinioni di tutti i Gruppi parlamentari presenti): quello della omogeneità della normativa su tutto il territorio nazionale, nel rispetto assoluto delle competenze delle Regioni e degli enti locali. Vi è la necessità che in tutto il territorio nazionale, e soprattutto nelle zone di interesse nazionale, quali sono le aree protette, siano siano stabiliti indirizzi che tutti devono seguire e ai quali tutti si devono uniformare e che possano quindi dare al cittadino un senso di certezza per quanto riguarda i suoi comportamenti in quelle zone. Voglio aggiungere, signor Presidente, onorevoli colleghi, che queste forme di intervento hanno anche un altro, profondo significato: quello

si rendano conto che quando si ragiona in termini di saggezza e di razionalità i comportamenti sono poi spontaneamente, e non obbligatoriamente, virtuosi. in questo che è un indirizzo con il quale ci vogliamo uniformare, sottolineo la facoltà per gli enti locali (in questo caso attraverso gli enti gestori per quanto riguarda le aree marine protette e per gli stessi enti locali laddove non

la responsabilizzazione delle popolazioni locali e la salvaguardia dell'ambiente rappresentano uno di quei passaggi essenziali perché le norme poi possano effettivamente trovare una positiva attuazione. Quindi, nel ringraziare nuovamente tutti, anche l'Assemblea del Senato per l'attenzione che ha voluto dedicare a questo provvedimento, ribadisco il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.